di esame del disegno di legge A.S. 2538, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno,

Signor Presidente, il disegno di legge in esame concerne la ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla messa al bando delle munizioni a grappolo ed è stato assunto quale testo base stante l'identità di materia con il disegno di legge n. 2321 già all'esame della Commissione medesima. Esso reca, peraltro, anche norme di adattamento dell'ordinamento interno. Ricordo in via preliminare che il Primo protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, contiene una serie di disposizioni che vietano gli attacchi militari indiscriminati a danno delle popolazioni civili e quelli realizzati con metodi o mezzi di combattimento che non sono diretti contro un obiettivo militare determinato. Le munizioni a grappolo (*cluster*), per le loro caratteristiche, rendono estremamente difficile rispettare le norme di diritto internazionale umanitario, previste a protezione delle popolazioni civili. Le *cluster* *bomb* sono infatti armi di grandi dimensioni che vengono sganciate da aerei o esplose da sistemi di artiglieria, in grado di rilasciare nell'aria bombe più piccole. Hanno una capacità di dispersione in un'area molto vasta e possono rimanere inesplose e colpire anche molti anni dopo. Un esempio degli effetti dell'utilizzo delle *cluster bomb* è quello registrato in Libano. In data 28 maggio 2008 l'Assemblea del Senato ha approvato all'unanimità un ordine del giorno che, raccogliendo le istanze contenute in alcune mozioni presentate da numerosi senatori,

giorno chiedeva al Governo italiano di assumere «nell'ambito della Conferenza di Dublino a seguito della dichiarazione di Oslo nel rispetto degli impegni internazionali nelle operazioni di pace delle Nazioni Unite, dell'Unione europea e dell'Alleanza anche in relazione alle esigenze di integrazione reciproca, una decisa posizione a favore della messa al bando delle *cluster bomb*» e «a sviluppare a tal fine un'adeguata iniziativa diplomatica per coinvolgere la comunità internazionale nell'adozione di uno strumento giuridicamente vincolante che proibisca la produzione e l'impiego di tali munizioni». La Conferenza di Dublino ha approvato il testo della Convenzione sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, aperta alla firma a Oslo il 3 dicembre successivo, che prevede la proibizione dell'uso, produzione, commercio e stoccaggio delle bombe a grappolo e impegna i Governi a distruggere gli *stock*, a bonificare i territori infestati e a fornire assistenza alle vittime. Ad oggi, la Convenzione di Oslo, è stata firmata da 108 Paesi, ratificata da 38, ed è entrata in vigore il 1° agosto 2010. Il segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon ne ha salutato con soddisfazione l'entrata in vigore. Il Governo italiano è stato tra i primi Paesi a firmare la Convenzione di Oslo lo stesso 3 dicembre 2008. Tuttavia, l'Italia non ha ancora provveduto alla ratifica. Quanto al disegno di legge, esso si compone di 8 articoli. Gli articoli 1 e 2 riguardano l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 prevede, al comma 1, la distruzione da parte del Ministero della difesa delle munizioni a grappolo e delle relative submunizioni esplosive. L'articolo 4 designa il Ministero degli affari esteri quale autorità competente per gli adempimenti previsti sul piano internazionale. I dati necessari al rapporto sono forniti dal Ministero della difesa e dal Ministero dello sviluppo economico. L'articolo 5 modifica la legge n. 58 del 7 marzo 2001 riguardante l'istituzione di un fondo per lo sminamento umanitario, prevedendo che le attività di bonifica comprendano anche territori con residui di munizioni a grappolo. L'articolo 6 stabilisce le condotte vietate relative all'impiego, alla produzione, all'acquisizione delle munizioni a grappolo e ne prevede le relative sanzioni. L'articolo 7 fornisce al provvedimento la necessaria copertura finanziaria spalmandone la spesa su cinque anni. L'articolo 8 prevede la deroga alla *vacatio*, in ragione della particolare urgenza che riveste la predisposizione dello strumento di ratifica della Convenzione. La Commissione, nel corso dell'esame del provvedimento, ha approvato alcuni emendamenti. È stato modificato il comma 3 dell'articolo 3 specificando che il mantenimento di una limitata quantità di armamenti è rinnovabile tramite trasferimento da altro Stato-parte. All'articolo 5 è stato inserito un comma aggiuntivo che precisa che l'attività di sensibilizzazione prevista dalla legge n. 58 del 2001 riguarda anche le munizioni a grappolo. È stato inserito un articolo aggiuntivo di modifica della legge n. 49 del 1987, includendo tra le attività di cooperazione con Paesi in via di sviluppo il sostegno e l'assistenza alle vittime delle mine antipersona e delle munizioni a grappolo. È stato poi modificato il comma 1 dell'articolo 6 nel senso che le sanzioni previste per l'impiego di bombe a grappolo siano estese anche a chi assiste finanziariamente tali attività.

agli articoli 5 e 8 e dell'ordine del giorno G8.100 di poter aggiungere ad essi la mia firma, perché ritengo siano delle necessarie integrazioni a questo disegno di legge di ratifica, che già ha subito, come ricordava poco fa il relatore, delle modifiche in sede di discussione in

non soltanto si parla di munizioni a grappolo ma anche di submunizioni a grappolo, e occorre insistere sulla necessità di articolare quanto più possibile gli obblighi relativamente a coloro che dispongono delle munizioni, dei diritti di brevetto e delle tecnologie idonee alla fabbricazione di munizioni a grappolo e submunizioni esplosive, oltre che naturalmente farci carico di quello che continua a essere uno dei problemi principali relativamente a tutti i nostri impegni, sia a livello nazionale che internazionale, e cioè la copertura finanziaria per poter dare adeguato seguito alle decisioni politiche che vengono prese. Sappiamo che sempre più spesso ci troviamo a dover ratificare dei trattati senza però essere in grado, dal punto di vista economico e finanziario, di darvi seguito o, ancora peggio, ci troviamo alle dei trattati (che, tra l'altro, portano il nome della nostra Capitale: penso, per esempio, allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale), salvo poi non prendere nessun tipo di di misura successiva per applicare o (con questo brutto neologismo che si usa oggi) implementare le norme ivi contenute. La ratifica di oggi è molto importante, e credo che ci possiamo prendere anche del tempo ulteriore approvando quegli emendamenti e anche l'ordine del giorno, anch'esso molto stringente, rimandando il testo alla Camera per un passaggio veloce. Penso non vi siano problemi e che, anzi, non soltanto un servizio utile all'idea che sottende a questo Trattato, ma si darebbe anche agli altri *partner* che fortunatamente sono stati più celeri di noi e hanno già ratificato questo Trattato facendolo entrare in vigore un esempio di come, in effetti, devono essere seguite le questioni. Ricordiamo che queste bombe continuano purtroppo a essere utilizzate in alcuni scenari dove oggi si usa la forza, e non perché si è in guerra, ma perché si ritiene di dover portare stabilità e sicurezza attraverso l'intervento militare. Credo però allo stesso tempo che ogni qualvolta ci si assume la responsabilità di utilizzare delle armi in un contesto in cui si porta la pace ci si debba assumere anche la responsabilità di eventuali errori, e questo lo lascio come spunto di dibattito: ogni volta si parla in casi come questo di trattati

nuova finestra"). Sono presenti in tribuna gli studenti dell'Istituto comprensivo «Angelo Casalini» di San Marzano di San Giuseppe, in provincia di Taranto. Rivolgiamo a loro il saluto del Senato e gli auguri per la loro attività di studio.

intervengo oggi molto volentieri in quest'Aula in un momento particolarmente significativo per il nostro Parlamento,

la mozione a prima firma della senatrice Pinotti, che poi confluì, insieme a quella del senatore Cantoni, in un unico atto, condiviso da tutti gli appartenenti al Senato.

potesse avvenire in tempi brevissimi, tanta era l'importanza dell'argomento affrontato e tanta era la condivisione da parte di tutti i parlamentari sulla soluzione che quelle due mozioni volevano conseguire. Ciò non è avvenuto, e purtroppo abbiamo dovuto attendere parecchio tempo. Oggi però siamo finalmente giunti alla fase finale di questo provvedimento. Il relatore ha già ricordato in maniera estremamente chiara ed incisiva cosa si intende quando si parla di bombe a grappolo. È una forma di minaccia che mantiene la sua pericolosità, la sua rischiosità nel tempo e che si traduce molto spesso in penalizzazioni, in sofferenze non tanto nei confronti del personale militare quanto nei confronti delle popolazioni che poi, dopo una crisi,

che l'Italia non poteva non accogliere con tutta la sua forza. La nostra Nazione è sempre stata, sotto questo aspetto, di esempio

il provvedimento che ci accingiamo a licenziare, credo sia opportuno sottolineare ancora una volta che il nostro Paese ha saputo evidenziare, anche in questo caso,

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo,

preliminare che il Primo protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, adottato l'8 giugno del 1977 e ratificato dall'Italia con legge 11 dicembre 1985 n. 762, vieta gli attacchi militari indiscriminati a danno delle popolazioni civili e quelli realizzati con metodi e mezzi di combattimento che non sono diretti contro un obiettivo Il medesimo Protocollo prevede la responsabilità di coloro che preparano o decidono un attacco, imponendo a questi ultimi di prendere tutte le precauzioni possibili nella scelta dei mezzi e metodi di attacco, allo scopo di evitare o quantomeno di ridurre al minimo il numero di vittime tra le popolazioni civili, nonché i danni ai beni di carattere civile che potrebbero essere incidentalmente causati. Le munizioni a grappolo, infatti, per le loro caratteristiche intrinseche, rendono quasi impossibile, o quantomeno altamente difficile, rispettare le norme di diritto internazionale umanitarie sopra richiamate, previste a protezione delle popolazioni civili.

Si tratta perciò di armi di grandissime dimensioni, sganciate da aerei o lanciate da sistemi di artiglieria, lanciarazzi e lanciamissili, in grado di rilasciare nell'area bombe più piccole. Si caratterizzano inoltre per la loro capacità di rimanere inesplose nel terreno e colpire anche dopo molti anni la loro dispersione, mantenendo inalterato nel tempo, purtroppo, il loro effetto letale.

evidenti gli effetti devastanti sulle ignare e inconsapevoli popolazioni civili. Il danno causato è immenso: si calcola che, delle 11.000 persone che ogni anno rimangono vittime di questi tremendi ordigni, il 98 per cento siano civili

che proibisce l'uso, la produzione, lo stoccaggio ed il trasferimento delle munizioni a grappolo, è stata approvata in occasione della Conferenza diplomatica di Dublino, firmata da 108 Paesi ed entrata in vigore il 1° agosto del 2010. La Convenzione impegna inoltre i Governi a distruggere gli *stock*, a bonificare i territori infestati e a fornire assistenza alle numerose vittime. L'Italia ha fornito un qualificato contributo al processo che ha condotto alla Convenzione sulle munizioni a grappolo, in linea con il tradizionale impegno del nostro Paese nel campo del disarmo. È vero che il Governo italiano è stato tra i primi a firmare la Convenzione di Oslo, precisamente il 3 dicembre 2008, ossia il giorno stesso dell'apertura alla firma; è però anche vero che, che, a distanza di più di due anni, l'Italia non ha ancora provveduto alla sua ratifica. Come sempre siamo in ritardo nel ratificare gli accordi stipulati, e come sempre siamo quindi causa di ritardo dei benefici che dagli accordi stessi potrebbero derivare. Non mi stancherò mai di dire che sarebbe opportuno dare attuazione immediata, ratificandoli, agli accordi che stiamo stipulando. Ritardare la ratifica di un accordo che proibisce l'uso, la produzione, lo stoccaggio e il trasferimento delle munizioni a grappolo, che causano danni intollerabili alle popolazioni civili è un atto grave. Non è più sopportabile l'uso dei mezzi bellici che vanno al di là delle necessità operative e causano inaccettabili danni alle popolazioni civili, e troppo spesso ai bambini. L'Italia dei Valori, ai bambini. L'Italia dei Valori, da sempre attenta alla tutela dei diritti umani, ritiene primaria l'importanza della ratifica della Convenzione in esame. È necessario infatti porre velocemente rimedio al grave ritardo del nostro Paese nella ratifica di questa Convenzione, che si caratterizza, tra l'altro, per un alto valore umanitario. Si tratta quindi di un provvedimento di notevole rilievo, una tappa fondamentale verso il disarmo mondiale per liberare il mondo da quelle che il Segretario generale della Nazioni Unite, Ban Ki-moon, ha definito armi ignobili.

Signor Presidente, il 1° agosto 2010 è entrata in vigore la Convenzione di Oslo che bandisce l'uso, la produzione, il trasferimento e l'accumulo delle munizioni a grappolo, che causano danni irrimediabili anche e soprattutto ai civili. È questo un grandissimo passo avanti sull'uso sconsiderato delle cosiddette bombe a frammentazione o a grappolo, che sono armi con sub-munizioni, ovvero bombe che contengono al loro interno decine di piccoli ordigni che si spargono sul terreno dopo l'impatto. Dal punto di vista umanitario, la problematicità di tali armi sta nella loro inaffidabilità: ciò, perché una percentuale delle munizioni lanciate non esplode al momento di colpire l'obiettivo, ma rimane sul terreno, trasformandosi in pericolosi residuati bellici esplosivi, che esplosivi, che causano vittime anche dopo la conclusione del conflitto. Infatti, una volta arrivate sul terreno, basta un nulla per farle esplodere, causando morti, mutilazioni e sofferenze non solo ai militari, ma anche e soprattutto alle popolazioni civili, e soprattutto ai bambini, che sono attratti dalla forma e dai colori di tali ordigni, costruiti apposta con malizia per essere motivo di attrazione. Ecco perché si può definire tale Convenzione un momento storico, un passo concreto e decisivo per porre fine a decenni di sofferenza di uomini, donne e bambini, con l'auspicio che la sua entrata in vigore influenzi e sproni a prendere una posizione anche quegli Stati che non vi hanno ancora aderito. Infatti, oltre a colmare una grave lacuna del diritto umanitario, l'accordo tende a dare una risposta forte e credibile ad un problema tuttora molto attuale. Lo stesso Santo Padre è intervenuto lo scorso 1° agosto sull'argomento, definendo tale disarmo un immenso passo avanti verso la tutela di quelle popolazioni sottoposte a bombardamenti, che si trovano alla mercé di uomini senza scrupoli che colpiscono indiscriminatamente bambini, ospedali e civili. La Santa Sede è stata inoltre tra le prime Parti a ratificare la Convenzione, nella certezza e nella consapevolezza che la logica della pace sia più forte della logica della guerra, che in tutti i casi deve avere come limite invalicabile la protezione e la tutela delle popolazioni civili ed in particolare delle persone più deboli e più vulnerabili. L'Italia ha fatto parte sin dall'inizio del primo gruppo di 46 Paesi che aderiscono alla Dichiarazione di Oslo sulle munizioni a grappolo e si è adoperata attivamente in seno alle riunioni ed alle conferenze preparatorie della riunione di Dublino del maggio 2008 alla definizione del testo finale di questo accordo. Signor Presidente, la ratifica all'ordine del giorno di oggi sancisce definitivamente la decisione italiana di mettere al bando questo tipo di armi, ponendo, oltre ai termini tecnici per il loro smaltimento, lo stanziamento economico per gli oneri complessivi relativi alle attività di distruzione delle scorte di munizioni di munizioni a grappolo in dotazione alle Forze armate italiane. Il nostro Gruppo ritiene che tale ratifica sia necessaria e di grande attualità. E' infatti ora di dire basta: basta alle notizie drammatiche che ci giungono ogni giorno dalle varie parti del mondo. Ormai da troppo tempo assistiamo inermi all'elenco di vittime civili, e soprattutto di bambini indifesi, vediamo popolazioni intere che a causa di questi ordigni disumani vivono ogni giorno in bilico tra la vita e la morte, inconsapevoli della subdola insidia che colpisce in maniera vigliacca ed indiscriminata e che fa e che fa arricchire anche uno sporco sistema di gente senza scrupoli che vive e lavora in funzione di un arricchimento personale. Per questi motivi, il nostro Gruppo esprimerà voto favorevole sul provvedimento in questione.

Presidente, con questo atto chiudiamo un percorso molto lungo, che parte dal 1949, all'indomani della Seconda guerra mondiale,

decidere di cambiare modo anche di combattere. Le regole che scaturiscono dalla Convenzione di Ginevra infatti obbligano tutti gli Stati ad adottare disposizioni per vietare attacchi militari indiscriminati che diano e che rechino danni esagerati alle popolazioni civili. Gli Stati sostanzialmente decidono che i Governi, o i decisori di attacchi, prendano in proprio la responsabilità e adottino precauzioni sulla scelta sia dei mezzi che dei metodi di attacco, per evitare al minimo i morti tra i civili. Oggi parliamo di un aspetto, di un tipo di munizionamento che riguarda le prescrizioni della Convenzione stessa: le famose *cluster bomb*, bombe a grappolo, che - è stato detto in più occasioni - sono ordigni, sì, di grandi dimensioni,

innanzitutto quello della bonifica di questi territori, perché nel tempo tutto si deteriora tranne che il potenziale esplosivo e dannoso di questi ordigni.

L'impegno che noi chiedevamo al nostro Governo di portare nella sede della comunità internazionale era che si vietasse sia l'uso, sia la produzione, sia la vendita,

Grazie,

efficacia militare - non portare mai attacchi indiscriminati che potessero mettere a repentaglio la vita dei civili. Questo è riconosciuto in tutti i teatri, non di guerra ma di presenza delle Forze armate e chi ha avuto modo di relazionarsi con le istituzioni e con le popolazioni locali non ha potuto che sentire parlare bene dell'approccio dei militari italiani. Anche questo, a onor del vero, va ricordato in questa occasione. finestra"). È presente in tribuna un secondo gruppo di studenti dell'Istituto comprensivo «Angelo Casalini» di San Marzano di San Giuseppe, in provincia di Taranto. Anche a loro rivolgiamo il saluto e gli auguri per la loro attività da parte del Senato.

penso che sia importante per l'Aula del Senato il fatto di essere giunti alla votazione di questa ratifica.

al di là delle dichiarazioni di intenti, non era mai arrivato ad un atto stringente. Ricordo, come hanno fatto alcuni colleghi, che uno dei primi atti

Si chiedeva al Governo, che di lì a poco, il 30 maggio, sarebbe andato alla conferenza di Dublino, di spingere il più possibile perché si arrivasse ad una volontà comune per la stipula di questa Convenzione e di impegnarsi poi direttamente

nell'approvare il disegno di legge sulle quote di genere nei consigli di amministrazione, si è ribadito come ci sia stata un'autonomia del Parlamento

una bella pagina di lavoro parlamentare. Credo che dovremmo ricordarlo, perché, come diceva il presidente Chiti, su temi che in realtà sono

tutte le Nazioni, soprattutto quelle che hanno più forza. Sono stati citati gli Stati Uniti, la Russia, quelle Nazioni che anche rispetto a questa Convenzione hanno ancora dei problemi; ebbene, ritengo ci debba essere una pressione internazionale perché si possa spingere il mondo a ragionare sul fatto che la violenza c'è, la guerra purtroppo è in atto, ma noi non possiamo assuefarci a questo, non possiamo accettare che si tratti di

e rimangono nel terreno per un tempo molto lungo, provocando un pericolo incredibile anche quando i conflitti sono terminati. terminati. Concludo questo mio intervento richiamando un'esperienza che ancora adesso mi emoziona molto quando la ricordo.

Grazie,

che è iniziata nel maggio 2008 con la Convenzione di Dublino ed aperta alla firma (e dunque sottoscritta dall'Italia e da altri 94 Paesi) nel dicembre dello stesso anno. Questa è una dimostrazione della volontà di intervenire su un settore che, come è già stato sottolineato, è estremamente delicato per la società nel suo complesso.

Voglio ringraziare il relatore, il Sottosegretario e tutti i colleghi delle Commissioni difesa e esteri che hanno messo testa e cuore in questa ratifica. Infatti, Infatti, la dimostrazione ce l'ha data l'Aula con una serie di votazioni praticamente all'unanimità. Le chiedo, signor Presidente, di poter lasciare agli atti il mio intervento,

il disegno di legge oggi al nostro esame, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, riguarda l'accordo con cui Italia e Slovenia consolidano la collaborazione e la mutua assistenza in ambito transfrontaliero, a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica...

L'Accordo integra precedenti atti pattizi intervenuti negli anni scorsi con la Slovenia, con particolare riferimento all'accordo tra i Ministeri dell'interno dei due Paesi nella lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e contro la criminalità organizzata, firmato a Roma il 28 maggio 1993, estendendo la cooperazione ad altri settori. Esso si inserisce nel più vasto contesto della collaborazione già in atto, a livello internazionale ed europeo, in materia di polizia, con particolare riferimento

L'Accordo individua le zone di frontiera ed indica gli organi competenti alla realizzazione dei citati obiettivi dell'articolo 1. I due Stati si impegnano ad informarsi reciprocamente sulle situazioni che possono comportare pregiudizi o comunque di interesse, sotto il profilo della sicurezza, effettuando periodicamente un'analisi congiunta degli aspetti che riguardano l'ambito transfrontaliero (articolo 2). I soggetti preposti all'applicazione dell'Accordo sono, per l'Italia, il Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, in qualità di organo centrale nazionale, e gli uffici periferici, nel quadro delle rispettive competenze; per la Slovenia, il Ministero dell'interno, la polizia, la Direzione generale di polizia in qualità di organo centrale nazionale con le proprie unità organizzative interne, nonché le unità organizzative di polizia di zona. Secondo i rispettivi ordinamenti nazionali, le richieste possono riguardare, tra l'altro, accertamenti in ordine ai proprietari e ai conducenti di veicoli stradali, di mezzi aerei e marittimi, alle patenti di guida, alle autorizzazioni relative al soggiorno, ai titolari di allacci telefonici o di altre apparecchiature di telecomunicazioni, all'identità delle persone e alla provenienza delle cose. Vengono altresì disciplinate disciplinate peculiari forme di cooperazione di polizia tra cui l'osservazione ed il pedinamento transfrontaliero nei confronti della persona indiziata di reato. È inoltre disciplinato l'istituto dell'inseguimento transfrontaliero, che può essere effettuato, nei casi d'urgenza, anche senza preventiva autorizzazione dell'altra parte contraente; quest'ultima può comunque chiederne l'interruzione immediata. La cooperazione tra gli organi di polizia riguarda, altresì, le operazioni di «consegne controllate» e le attività sotto copertura, che le parti si impegnano ad agevolare. L'Accordo prevede un'adeguata tutela per la trattazione delle informazioni e dei dati sensibili ed è infine sancita la possibilità di respingere, anche parzialmente, le richieste di collaborazione, qualora esse possano compromettere la sovranità, la sicurezza, la legislazione nazionale od altri interessi primari. Gli oneri dell'attuazione dell'Accordo sono stimati solo in 93.610 euro, a decorrere da quest'anno. Vorrei richiamare la mia esperienza con l'Organizzazione della cooperazione e la sicurezza in Europa, dalla quale è emersa con chiarezza l'importanza della tutela della frontiera italo-slovena in un'ottica di contrasto all'immigrazione clandestina, che ho personalmente vissuto per diversi anni, quando abitavo lì. Sottolineo altresì la necessità di mantenere ed incrementare le relazioni bilaterali tra i due Paesi. In conclusione, la Commissione propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo».

sull'Atto Senato n. 2524 di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia. L'Accordo oggetto della presente ratifica è reputato da me e dal Gruppo dell'Italia dei Valori di estrema importanza. Un Accordo con cui l'Italia e la Slovenia consolidano la collaborazione e la mutua assistenza in ambito transfrontaliero, a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Si tratta di un provvedimento, colleghi, di notevole rilevanza anche al fine di meglio potenziare l'attività di contrasto alla criminalità organizzata internazionale. L'Accordo va ad integrare i precedenti atti pattizi intervenuti negli anni scorsi con la Slovenia e si inserisce nel più ampio contesto della cooperazione già in atto a livello internazionale ed europeo in materia di polizia, con particolare riferimento alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen. L'Italia e la Slovenia, anche attraverso questo Accordo, si avvicinano e rafforzano il loro rapporto. In un mondo ormai globalizzato è importante che anche i Paesi più piccoli si accordino nell'interesse della sicurezza dei cittadini. Ritengo quindi che si tratti di un provvedimento di importanza strategica a tutela della sicurezza di entrambi i Paesi. Signor Presidente, colleghi, prima di concludere, desidero sottolineare come l'Accordo che stiamo ratificando oggi è stato firmato già nell'agosto del 2007, e la Slovenia, un piccolo Paese, lo ha ratificato esattamente a ottobre 2007. Ecco noi,

Sarebbe opportuno, infatti, dare attuazione immediata, ratificandoli, agli Accordi che vengono stipulati come ha fatto, ripeto, la Slovenia. Per questi motivi,

anche con me stesso, perché non riusciamo a far capire a queste persone - chiamiamole così e mi scuso se vi qualifico persone - che questi sono atti importanti, come quelli precedenti, ma vedo che l'ignoranza regna sovrana per questi argomenti.

Uno che è senz'altro vero, è che il senatore Pedica ha usato espressioni che non sono corrette e non sono rispettose

Per favore, lei dovrebbe essere richiamato ogni tre secondi: ha fatto di quel banco un centro di biblioteca dove si viene a leggere i giornali! Capisco il suo sforzo sociale, ma non esageriamo!

un momento di attenzione, mentre quando c'è attenzione anche senza scontro si producono gli atti più positivi e provvedimenti che hanno un senso, come stamani. E questo è un errore che compiamo tutti, ed è giusto che non vi sia, perché c'è un rispetto e un decoro per l'Aula.

sottolineare come questa ratifica sia fortemente richiesta dalle istituzioni della Provincia di Gorizia, prefettura e questura in testa, che anche in una nostra recente visita come Comitato Schengen hanno sollecitato

sulla cooperazione transfrontaliera di polizia stipulato a Lubiana il 27 agosto 2007. Va sottolineato come la Slovenia abbia ratificato l'accordo nello stesso anno, a dimostrazione che c'è da parte dello Stato contraente vivo interesse per la collaborazione con il nostro Paese. Voteremo a favore del disegno di legge n. 2524 di ratifica e di esecuzione dello stesso per diversi motivi che cercherò, brevemente di illustrare. La nostra posizione è motivata da una duplice valutazione: una di carattere prettamente tecnico e riguarda i contenuti del provvedimento e le ripercussioni positive sulla comunità e l'altro di carattere più generale e politico rispetto agli importanti progressi fatti negli ultimi tempi nei rapporti tra l'Italia e la Slovenia. Slovenia. A questo proposito vorrei sottolineare che la ratifica avviene in un momento di grande vivacità nelle relazioni tra i due Paesi. Quanta strada è stata fatta da quel lontano 1981, anno in cui si è svolta la prima edizione della manifestazione «confine aperto - Odprta meja» nel comune di Dolina San Dorligo Della Valle di cui domenica prossima celebreremo insieme il trentesimo anniversario. Dal punto di vista degli scambi commerciali l'Italia risulta essere il secondo Paese fornitore e cliente della Slovenia dopo la Germania.

che ha segnato un punto di eccellenza nel processo di rafforzamento dell'amicizia tra l'Italia e la Slovenia. Recentemente è stata anche costituita l'Associazione interparlamentare di amicizia con Slovenia, a cui hanno aderito oltre 70 deputati e senatori di tutti gli schieramenti politici e della quale mi onoro di essere Presidente. Un'analoga associazione di amicizia con l'Italia si è costituita ancora prima presso il Parlamento di Lubiana e in breve ci sarà qui a Roma un incontro bilaterale. È anche importante che questo provvedimento sia stato approvato sia alla Camera che in Commissione affari esteri del Senato all'unanimità. Si tratta certamente di piccoli gesti, ma comunque impensabili solamente qualche anno fa, a dimostrazione che il clima è veramente cambiato e tutta l'area transfrontaliera, storicamente caratterizzata dalla presenza di lingue e culture diverse, al contempo penalizzata nel passato dalla "cortina di ferro", ha oggi davanti a sé grandi opportunità. In questa direzione va anche l'Accordo di cooperazione transfrontaliera di polizia che risponde all'esigenza di rafforzare la collaborazione bilaterale in materia di sicurezza e si propone di potenziare l'attività di contrasto alla criminalità organizzata internazionale e all'immigrazione clandestina. Tutto ciò produce vantaggi per la collettività in relazione ad una più elevata qualità dei controlli a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Non mi dilungherò sui singoli articoli. Desidero solo sottolineare si tratta di alcuni strumenti molto importanti e innovativi: dalla previsione della collaborazione nel campo della formazione, alla possibilità di istituire gruppi di lavoro e di indagini miste, al distacco temporaneo di funzionari per lo svolgimento di attività di sostegno e consultazione, alla possibilità del pattugliamento misto lungo il confine di Stato,

che negli ultimi tempi sono in parte diminuiti i flussi di criminalità organizzata e di immigrazione clandestina attraverso il confine mi sembra di poter affermare che questo si accompagna al progredire del processo di avvicinamento dei singoli Paesi all'Unione europea. Accelerando l'integrazione si contribuisce anche alla stabilizzazione, alla diminuzione della criminalità, alla legalità. Anche per questo chiediamo al Governo di assumere un ruolo più incisivo in quell'area, un impegno più forte rispetto a questo tema nell'ambito europeo. Un ultimo rilievo: penso che questo Accordo vada implementato ed arricchito con ulteriori Accordi di collaborazione in tema di sicurezza. Alcune importanti iniziative sono già operative. Mi riferisco ad esempio alle esercitazioni comuni delle forze militari, come anche all'Accordo a livello regionale sulla collaborazione della Protezione civile in caso di incendi o altre calamità naturali. Tutto ciò va certamente a beneficio della popolazione locale, che è stata nel passato penalizzata ed emarginata, Ma l'Accordo che oggi ci apprestiamo a ratificare riguarda complessivamente l'Italia e la Slovenia, alle quali apre nuovi orizzonti di collaborazione, di amicizia e di impegno comune per un futuro di pace e di sviluppo. Per tutte le ragioni che ho cercato di illustrare il Gruppo del Partito Democratico voterà convintamente il disegno di legge di ratifica dell'Accordo. *(CN)*. Signor Presidente, il disegno di legge n. 2524 riguarda l'Accordo con cui l'Italia e la Slovenia consolidano la collaborazione e la mutua assistenza in ambito transfrontaliero,

Il relatore, senatore Azzollini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi

al nostro esame che, come è noto, è un provvedimento di sistema (se così posso dire), cioè un atto che incide strutturalmente sul bilancio dello Stato e, direi di più, sulla manovra economica che di anno in anno il Governo ha necessità di proporre al Parlamento. Nella Commissione bilancio sono stati affrontati punti decisivi, anche e soprattutto in rapporto alla *governance*

oggetto di attenzione da parte della Commissione bilancio. Su sollecitazione anche dei colleghi dell'opposizione, abbiamo preso posizione su tali questioni

nuove linee guida che l'Unione europea si appresta a dare agli Stati membri proprio nella costruzione dei bilanci. Sul piano tecnico si chiameranno modifiche del Patto di stabilità, linee di *governance,* ma di fatto vi è una connessione tra queste grandi questioni e la costruzione del bilancio.

legati essenzialmente al fatto che il semestre europeo che parte quest'anno e che rappresenta un assetto a regime del coordinamento in materia economica all'interno dell'Unione europea comporta un ripensamento delle scadenze del ciclo della programmazione nazionale. Essenzialmente il primo obiettivo del testo approvato dalla Camera dei deputati è quello di anticipare al 10 aprile la presentazione del documento programmatico di finanza pubblica, da approvare da parte del Parlamento entro la fino dello stesso mese per fornire alla Commissione europea il quadro degli obiettivi che il nostro Paese si propone. Seguono poi la procedura di assegnazione a ciascun Paese dell'entità delle varie manovre e la successiva sessione di bilancio. Sempre tenendo conto delle richieste europee, si è dovuto poi ristrutturare il documento programmatico per tener conto non solo di tutte le affermazioni e degli elementi relativi alla finanza pubblica, ma anche per far approvare al nostro Paese il Programma nazionale di riforma di cui devono essere enunciati i principali contenuti nelle stesso documento programmatico. Tutto questo ha anche implicato una rivisitazione delle modalità di coinvolgimento delle autonomie territoriali, nonché una diversa strutturazione della Nota di aggiornamento, da presentare a settembre, confinata alla modifica delle previsioni, fermi rimanendo quindi gli obiettivi fissati a aprile, così come eventualmente aggiornati, essenzialmente sulla base delle decisioni comunitarie. Al di fuori di quest'ultima ipotesi, quindi, il nostro Paese si adegua in sostanza all'impostazione europea di variare l'entità delle manovre con oscillazioni delle previsioni, ma tenendo fermi gli obiettivi. Un altro passaggio di rilevo del testo è che si consente, con la legge di stabilità, di iscrivere nuovi oneri correnti con copertura sul miglioramento del risparmio pubblico solo se si tratta di riduzioni di entrata. Un incremento della spesa corrente, quindi, per esempio effettuata con le tabelle della legge di stabilità, deve trovare coperture con mezzi presenti nello stesso disegno di legge di stabilità e non può più attingere dunque alle maggiori risorse provenienti da un migliore andamento a legislazione vigente. Va sottolineato con forza che ciò spinge, a parità di condizioni, verso una minore crescita della nuova spesa, con un meccanismo che si colloca in pieno nell'alveo degli indirizzi europei volti a ridurre il tasso di crescita della spesa pubblica. Se si combina questa innovazione con l'altra secondo cui tutte le maggiori entrate rispetto alle previsioni non possono essere utilizzate a copertura e quindi devono essere devolute a beneficio del *deficit*, si comprende come anche sotto questo aspetto il nostro Paese recepisce in pieno l'indirizzo comunitario, nel senso di contenere la spesa e soprattutto di incidere sul debito. Non utilizzare tali entrate significa infatti ridurre il *deficit* e quindi rallentare la formazione di nuovo debito. Per usare una parola che è stata oggetto per lunghi anni di tante campagne, si può dire che non è più possibile, quindi, utilizzare eventuali tesoretti. Va poi sottolineato che si accentua il momento programmatico estendendo anche sulle spese non rimodulabili la tecnica della programmazione triennale, il che rappresenta un terzo elemento positivo in termini di uno strumento aggiuntivo di controllo sul medio periodo dell'evoluzione della spesa. A questo ultimo riguardo, opportunamente, il testo prevede che comunque l'adozione della tecnica della fissazione di limiti pluriennali per le spese di bilancio debba comunque tener conto delle peculiarità delle spese non rimodulabili. Si tratta di una previsione improntata a grande realismo perché consente al Governo di evitare un critico automatismo nella definizione di tetti di spesa quando si tratta della gran parte della spesa dello Stato di natura obbligatoria e inderogabile. Poiché è da verificare che tutta questa spesa, che supera il 90 per cento del totale, possa essere gestita con tecniche automatiche, che calino dall'alto limiti che si possono poi rivelare nel corso del tempo come insostenibili sul piano non solo tecnico, ma anche e soprattutto politico-sociale, l'articolazione del testo consente quella flessibilità necessaria per tener conto delle varie tipologie e situazioni. In proposito ricordo che vi fu un momento in cui era in auge il cosiddetto metodo Gordon Brown, i cui

Come quarto elemento di novità sotto il profilo dell'accresciuto impegno del nostro Paese per concorrere a realizzare gli obiettivi comunitari in materia di controllo della finanza pubblica e riduzione del debito, va menzionato che la prima sezione del DEF accentua l'obbligo di esplicitare gli obiettivi di accelerazione di tale riduzione, con ciò dando il giusto e prioritario rilievo alla necessità di dare corso alle indicazioni europee. Per quanto riguarda il lavoro svolto in Commissione (da qui la necessaria premessa), si sono discusse numerose ed importanti questioni.

da parte delle pubbliche amministrazioni abbandonare il sistema della competenza, dopo quasi un secolo di sua validità, e lasciare che i conti venissero espressi e gestiti solo in termini di cassa. Ferma rimanendo l'importanza di rilanciare la cassa, sulla base sia delle indicazioni europee sia del fatto che questa contabilità permette di cogliere nel migliore dei modi l'impatto sull'economia dell'operatore pubblico, si è affinata, con un apposito emendamento approvato in Commissione, la delega relativa al potenziamento di tale profilo, ma si è al contempo prevista anche una delega di semplificazione e di maggiore trasparenza della parte relativa alla competenza. Il sistema sembra più equilibrato, ovviamente nell'intesa

Un altro punto su cui si è intervenuti in Commissione riguarda la semplificazione delle modalità di coinvolgimento delle autonomie nella fase di decisione della programmazione finanziaria annuale di medio periodo. Il testo che ci perveniva dall'altro ramo del Parlamento è sembrato troppo complicato nei passaggi procedurali, e la soluzione che è stata votata prevede che le autonomie vengano coinvolte esprimendo un parere sul documento del Governo in tempo utile perché le Camere possano approvare il documento stesso, da inviare poi all'Unione europea. Con un altro emendamento è stata colta l'esigenza di evitare che i provvedimenti collegati, per i quali non esiste più un termine massimo di presentazione al Parlamento, sulla base del testo pervenutoci dalla Camera, fossero tali da ricreare la figura del "collegato" di sessione, tale quindi da entrare nella definizione dei saldi. Ne consegue che con questa specificazione si è inteso far rimanere il collegamento tra questa figura di provvedimento e la strategia di sviluppo che il Governo intenda varare. Un altro blocco di questioni ha riguardato la soluzione di alcuni problemi che si stanno ponendo per quanto riguarda l'operatività dell'ISTAT.

Altra questione affrontata è quella della Relazione generale sulla situazione economica del Paese: anche qui si è effettuata un'opera di semplificazione, nel senso di prevedere una commissione, a cui partecipa l'ISTAT, che nel giro di due mesi propone forme di ristrutturazione del contenuto di questo documento, la cui presentazione per il 2011 rimane quindi al 30 settembre, fermo rimanendo che a regime essa è fissata al 30 aprile. Altre questioni sono state affrontate e verranno riprese qui in Assemblea quando si tratterà di discutere i singoli emendamenti, che a mio avviso saranno oggetto dell'intervento del collega di opposizione, per cui è più

Per intanto, mi preme sottolineare che in definitiva, sia pure sotto l'incalzare degli stimoli provenienti dall'Europa, si sono colti tre obiettivi di fondo. Anzitutto, si è allungato e irrobustito il criterio della programmazione a medio termine; in secondo luogo, si sono previsti istituti che sostanziano un maggior coinvolgimento del Parlamento nella definizione di questi obiettivi; in terzo luogo, si è stabilito un collegamento tra le politiche congiunturali e di coordinamento macroeconomico da un lato, e la politica delle riforme Il tutto, con un coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche non statali. Con tale provvedimento, l'Italia è uno dei Paesi che ha modificato più velocemente le proprie normative contabili per tener conto delle decisioni europee, il che contribuisce a dare credibilità,

e per la definizione della programmazione economica, le innovazioni necessarie a renderla coerente con le nuove regole adottate dall'Unione europea. Una discussione seria su questo tema si può però sviluppare solo dopo che si sia risolta una vera e propria questione preliminare, che Noi, la politica italiana, il Governo, la maggioranza, l'opposizione, partecipiamo alla discussione che è in corso nell'Unione europea sulle regole, le procedure, i contenuti e gli obiettivi del coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri con l'obiettivo esclusivo, comunque prevalente, di mitigare l'impatto sul nostro sistema nazionale delle decisioni che verranno prese? Oppure vi partecipiamo con lo scopo ambizioso e dichiarato di affrontare le cause che hanno condotto al fallimento del Patto di stabilità e crescita, all'incapacità di governare gli squilibri macroeconomici dell'area dell'euro e che, per questa via, hanno messo a rischio l'esistenza stessa della moneta unica? Non si può - questa è la mia opinione - stare da protagonisti nel confronto aperto se prima non si risponde con precisione a tale domanda. Se la risposta è la prima, il nostro obiettivo si traduce in Europa nel chiedere uno sconto. Questo, in sostanza, il discorso che implicitamente rivolgiamo ai nostri *partner* europei: sì, voi volete regole più rigorose sul *deficit* e sul debito, e noi le approviamo, anche se, dipendesse da noi, ne faremmo volentieri a meno, ma vi chiediamo di applicarcele con moderazione considerando che, se è vero che abbiamo un debito pubblico molto alto, è altrettanto vero che il settore privato dell'economia (in particolare le famiglie) è decisamente meno indebitato rispetto a quello di altri Paesi. In Italia questo approccio, che chiamerò minimalista, induce invece a minimizzare. Questo è il discorso che implicitamente in quel caso rivolgiamo al nostro Paese: c'è il nuovo Patto di stabilità, e per noi rispettare le nuove regole sarà difficile, ma non è cosa di oggi, poiché se ne parla dal 2014. Quante volte il Ministro dell'economia e delle finanze ha già ripetuto questa frase? non potrà esserci vero rigore alla dimensione europea perché ci sono altri che stanno peggio di noi, e non solo tra i Paesi periferici: avete presente quanti titoli di debito sovrano a rischio hanno nel loro attivo le grandi banche della vecchia area del marco? Avete visto a che livello è giunto nel 2010 l'indebitamento strutturale della Francia? Tutto l'opposto se scegliamo invece la seconda strada. Questo è il discorso che potremmo esplicitamente rivolgere ai *partner* europei e al nostro Paese nel Consiglio europeo del 24 e 25 marzo

di evoluzione della spesa, di riduzione dell'indebitamento strutturale e di riduzione in tempi certi del volume globale del debito pubblico. Ora siamo qui, in Europa, forti delle nostre potenzialità e consapevoli dei nostri limiti, per costruire insieme a voi regole politiche comuni per la stabilità, la crescita e la coesione sociale e proponiamo un nuovo salto nella costruzione del mercato unico secondo le proposte del rapporto Monti. Proponiamo la gestione comune, sul merito di credito dell'Europa e non di ogni singolo Paese, di quote del debito sovrano proporzionali al prodotto; proponiamo investimenti in infrastrutture materiali e immateriali, *in primis* l'interconnessione delle grandi reti energetiche, per la ricerca scientifica e per l'innovazione, finanziati tramite l'emissione di *eurobond*, come il nostro Ministro dell'economia ha recentemente riproposto assieme al presidente dell'Eurogruppo Juncker. Proponiamo politiche fiscali a dimensione europea volte a disincentivare la speculazione a breve e a ridurre le dimensioni della leva finanziaria degli istituti di credito».

Naturalmente, potevamo fare diversamente: potevamo burocraticamente sederci sopra i risultati raggiunti dalla Camera, a mio giudizio perfettamente insoddisfacenti. Gli emendamenti che abbiamo presentato, e che riproponiamo per l'Assemblea, discendono con coerenza da questa ispirazione, che si può condividere o no, ma è e rappresenta il fulcro di una scelta fondamentale per il futuro dell'Italia nei prossimi decenni, non nei prossimi mesi. Il Governo e la maggioranza hanno respinto questa proposta, un po' perché, penso, non vogliono, e molto perché non ritengono di potere, di avere la forza politica necessaria per una scelta così impegnativa. Ma noi non perdiamo la fiducia nel nostro potere di persuasione, e quindi insistiamo sulla nostra proposta. Cercherò ora di riassumerne i cardini essenziali, e procederò per punti, con l'obiettivo di rendere chiaro che ciò che proponiamo di scrivere nella nostra legge di contabilità non pretende di anticipare ciò che sarà deciso in termini di nuove regole dal Consiglio europeo del 24 e 25 marzo: la regola che proponiamo di adottare nella nostra proposta fondamentale è riassuntiva di una strategia di riequilibrio e stabilizzazione della finanza pubblica che sarebbe indispensabile adottare, secondo noi, *etsi Europa non daretur*, anche se l'Europa non ci fosse, e nella nella consapevolezza che, adottandola, in Europa peseremmo di più e ci presenteremmo con una più forte credibilità, e dunque con maggiori possibilità di costruire consenso su proposte, come quella a favore degli *eurobond*, che uniscono in Italia maggioranza e opposizione. Di qui la proposta fondamentale che abbiamo avanzato: scrivere ora, adesso, nella legge di contabilità, prima del 24 e 25 marzo, una regola di miglioramento del saldo che ci conduca al pareggio strutturale nel 2017.

non ha atteso le decisioni europee; anzi, ha scelto di agire autonomamente, anche perché pensa di influenzare per questa via le decisioni europee. È ciò che si definisce, nel caso della Germania, ambizione egemonica: legittima ambizione egemonica. La ragione per la quale noi non facciamo altrettanto non è che "non possiamo permettercelo", come qualcuno dice. Tremonti ha ragione quando rivendica le nostre ragioni di forza. Le ha elencate tante volte, e io stesso le ho richiamate. Ma è adesso che si dimostra se dietro questa legittima rivendicazione delle nostre ragioni di forza c'è una razionale strategia e una grande ambizione politica, o solo il tentativo di "passare la nottata" e una debole propaganda. Primo punto. L'OCSE da tempo raccomanda che la decisione di bilancio annuale - su questo, il testo che viene dalla Camera è utile - venga preceduta dall'approvazione di un documento con un orizzonte temporale molto più lungo: almeno, come si dice in termine tecnico, un obiettivo di medio termine. Questa esigenza, presente ovunque, è più forte nei Paesi che manifestano rilevanti squilibri di finanza pubblica. Noi, purtroppo, siamo tra questi. E non da oggi, non dalla grande recessione. Secondo punto. Le regole fiscali europee hanno subito nel tempo delle revisioni molto profonde. In particolare, nel 2005 - non ieri mattina per rendere il Patto meno "stupido" - come diceva il presidente della Commissione Prodi - si decise che il limite di *deficit* del 3 per cento valesse per il saldo strutturale, e non più per quello nominale. Obiettivo di questa iniziativa era rendere il Patto più flessibile, meno stupido, meno prociclico, come si dice in termine tecnico. Più margini per politiche fiscali espansive in tempi cattivi, in cambio di maggiore rigore nei tempi buoni dello sviluppo economico. Cos'è, infatti, il saldo strutturale? È il saldo di bilancio corretto per il ciclo. Definito, cioè, il saldo nominale di bilancio, è possibile correggerlo facendo emergere il peso esercitato dall'andamento del ciclo economico nel determinare il saldo stesso.

Quarto punto. Con la grande recessione e la successiva crisi dell'euro, è emersa l'insufficienza del Patto di stabilità e crescita. la decisione, già assunta, di rivederlo: nuovo Patto di stabilità e crescita, nuova attività di coordinamento, semestre europeo e programma nazionale delle riforme. Cosa ci si propone di raggiungere, con questa revisione? Fondamentalmente due cose: mantenere l'obiettivo di medio termine e la strategia del miglioramento dello 0,5 per cento del saldo strutturale fino al raggiungimento del pareggio strutturale,

In particolare, nei Paesi che hanno già conseguito l'obiettivo di medio termine, la spesa non deve crescere più del tasso di crescita "prudente" del PIL, termine che significa previsto in modo prudenziale nel medio e lungo termine. termine. I Paesi che non hanno conseguito l'obiettivo di medio termine devono avere un tasso di crescita della spesa inferiore al tasso "prudente" di crescita del prodotto.

Quinto punto. Tutto ciò non è aria fritta, non è roba per tecnici: tutto ciò è la sostanza della politica. L'adozione di questa regola sull'obiettivo di medio termine e sulla spesa implica che il suo mancato rispetto dia luogo: all'avvertimento da parte della Commissione, poi alla raccomandazione da parte del Consiglio e, quindi, alle sanzioni. Sesto punto.

La proposta della Commissione - adesso sappiamo che il 24 e il 25 marzo verrà adottata - è la seguente: ogni anno un ventesimo di miglioramento del debito in meno della differenza tra debito raggiunto - in Italia sostanzialmente il Per noi la differenza è 60 (120 meno 60) e un ventesimo di 60 è 3: sono 45 miliardi di debito in meno ogni anno. le due regole non si elidono, ma si sommano. La regola sull'indebitamento strutturale e sulla evoluzione della spesa si somma a quella sul debito. È tuttavia molto interessante notare che uno scrupoloso rispetto della prima regola, quella sull'indebitamento strutturale, che noi proponiamo di adottare nella legge di contabilità,

Secondo Ignazio Visco della Banca d'Italia e secondo lo studio del Servizio del bilancio del Senato - come al solito particolarmente accurato, e di questo lo ringrazio assumendo una crescita costante del PIL del 2 per cento di qui al 2020, il pareggio strutturale (ossia l'obiettivo di medio termine) verrebbe raggiunto nel 2017. Quando si parla di questi problemi, vuol dire domani mattina. Già nel 2020 il debito cadrebbe sotto cento del prodotto, per raggiungere il 60 per cento - ossia l'obiettivo di Maastricht - nel 2037; e questo solo rispettando la regola - intendiamoci, molto impegnativa - dell'indebitamento strutturale che migliora fino al pareggio nel 2017. Settimo punto. Naturalmente, in quale fase si concentrano le difficoltà di questa scelta politica? Nei primi anni, dal 2011 al 2017, perché il rapporto tra spesa e prodotto dovrebbe avere questo andamento. Bisogna saperlo, e noi che proponiamo questa regola lo sappiamo, non siamo utili idioti: sappiamo che adottare quella proposta significa trarre queste conseguenze. In primo luogo, la spesa pubblica non dovrebbe crescere per nulla da qui al 2017. In secondo luogo, dopo il 2017, la spesa potrebbe tornare a crescere, ma non più del prodotto stimato prudentemente. Ottavo punto. Queste regole sull'indebitamento strutturale sono già parte dei vincoli determinati dalle scelte europee. Le regole sulla spesa saranno invece ulteriori e saranno sicuramente adottate, perché servono per rendere credibili le decisioni già prese a proposito dell'obiettivo di medio termine. E abbiamo poi visto che la regola sul debito - ne ho appena parlato - ci vincola a scelte analoghe o identiche. Ma anche se il 24 e il 25 marzo andasse male - Dio non voglia, per l'euro facesse l'accordo, possiamo dare per certo che non verrà comunque indebolito il Patto di stabilità e crescita, così come ridefinito nel 2005. Anzi, è probabile che qualche elemento di rafforzamento ci sarà. Nono e conclusivo punto. Berlusconi e Bossi, i due *leader* della coalizione di Governo, hanno deciso di "andare avanti", per usare la loro espressione. Hanno rinunciato - o sono stati costretti dalla loro crisi a rinunciare - a giocare la carta del ricorso anticipato alle urne. Ne prendiamo atto. La domanda cui essi debbono però rispondere è semplice e immediata: vanno avanti per tirare stancamente e disperatamente a campare, o vanno avanti per imporre al Paese il cambiamento che pure proclamano di ritenere necessario? Misurata sulle scelte compiute in tema di regole di gestione della finanza pubblica e di nuova *governance* economica europea, la risposta, purtroppo, è inequivocabile: cercano di tirare a campare. Compete dunque a noi, al principale partito di opposizione, asse dell'alternativa di governo, mostrare fiducia nel Paese e lanciare una sfida per il suo rilancio: se il Governo la raccoglie - come io mi auguro ancora, nel corso di questo dibattito in Aula - tanto meglio, per il Paese e per noi; se la respinge - come ha fatto fino ad oggi - darà esso stesso la prova più limpida della sua - insopportabile, ormai! - inadeguatezza.